è convocato per domani, mercoledì 24 ottobre, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale». Voteranno per primi i deputati.

Vorrei evidenziare alcune notizie arrivate ieri, grazie anche all'impegno di SOS Impresa, l'associazione diffusa nel territorio che aiuta i commercianti a denunciare il *racket* e le estorsioni. Qualcuno si è anche lamentato del fatto che i giornali, in questo giorno, potessero dedicare grande spazio

sarebbe oggetto di pressioni anomale da parte del banchiere Profumo per impedire una sua eventuale candidatura alla Presidenza della Sempre nei giorni scorsi, su tutta la stampa nazionale, abbiamo letto che il professor Bazoli ha inviato una lettera al direttore del «Corriere della Sera» Paolo Mieli per richiamarlo alla ortodossia ulivista. Presidente,

tenta di impedire una candidatura alla Presidenza di una Regione e un altro banchiere, con una lettera al direttore del «Corriere della Sera», cerca di imporre un mutamento di linea politica. Questo, secondo me, signor Presidente, è un vero e proprio squadrismo bancario, di quei poteri forti che sostengono questo Governo. Ecco perché le chiedo di fare chiarezza

necessiti di un'attenzione giornaliera da parte del Governo e, quindi, saluto positivamente il fatto che oggi il Governo è riunito per varare il pacchetto sicurezza che anche in Commissione antimafia abbiamo sollecitato.

denunce. Si sono manifestati segnali fondamentali e positivi che riguardano anche le scelte delle grandi strutture che difendono gli interessi delle imprese.

il fenomeno della cosiddetta collusione partecipata. In Sicilia si parla di imprese legate alla cosiddetta borghesia mafiosa. Quando inizialmente gli appalti venivano gestiti

Molto spesso queste imprese sono state obbligate volutamente e in maniera connivente a pagare le estorsioni. È un metodo che bisogna assolutamente debellare. In Sicilia è capitato con gli industriali vinicoli, che hanno assunto

per smetterla di assistere a questo aspetto della questione meridionale. Va detto a tutti gli amministratori del Sud e a coloro che in questo momento gestiscono la cosa pubblica. In Sicilia le risorse europee non sono assolutamente servite a far fare un salto di qualità né all'economia

mettendo in evidenza alcuni aspetti di carattere generale che ritengo importanti per per affrontare questa discussione, riguardante un provvedimento al quale sia il Governo, sia la maggioranza assegnano un'importanza particolare. Il provvedimento si inserisce nella politica economica generale del Governo e gli obiettivi globali sono il risanamento, l'equità e lo sviluppo.

e, in particolare, dalla lotta all'evasione, che ha prodotto risultati importanti dal punto di vista delle entrate fiscali. è un recupero della base imponibile e si inizia - attraverso alcune iniziative, come anche questo provvedimento - la restituzione progressiva nei confronti dei contribuenti.

Presidente, la ringrazio. Dicevo che il provvedimento è possibile grazie al fatto che la lotta all'evasione ha prodotto risultati importanti: vi è un recupero della base imponibile e si inizia a restituire ai contribuenti, con un'azione progressiva nei loro confronti, per poter intervenire, appunto, con azioni di equità e di redistribuzione sociale.

Mi auguro che la finanziaria che esamineremo nei prossimi giorni riesca a garantire la copertura non solo per il 2007, come previsto dal decreto, ma anche per gli anni a venire, rendendo strutturale l'iniziativa relativa alla quattordicesima per le pensioni basse. La copertura è prevista anche con l'utilizzo di una parte del FAS (il Fondo per le aree sottoutilizzate):

al Sud, in particolare per quanto riguarda gli investimenti delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS, la maggior parte degli interventi nelle infrastrutture.

le misure a favore degli incapienti, il finanziamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia, i trasporti per migliorare il servizio metropolitano e ferroviario e il settore della scuola. C'è inoltre un'iniziativa molto importante che riguarda il ripristino dei contributi agli organismi internazionali per la pace e gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo per 910 milioni. Vi sono inoltre anticipazioni di risorse per il rinnovo del contratto del pubblico impiego per un miliardo di euro. Queste iniziative denotano, quindi, il carattere sociale del provvedimento.

Più nel dettaglio, voglio ricordare il cosiddetto piano‑casa, cui complessivamente sono destinati 700 milioni di euro, finalizzati al recupero di alloggi ex IACP o dei Comuni, all'acquisto, all'affitto e alla costruzione di alloggi da destinare agli sfrattati. Vi sono inoltre misure importanti di grande valore sociale. Certamente

un tetto di spesa; quindi, si potrebbero ingenerare alcuni problemi dal punto di vista dell'accessibilità di coloro che potrebbero essere interessati da questa norma. Inoltre, è solo per quest'anno: non è ancora una norma, per così dire, permanente. Auguriamoci che nei prossimi anni si riescano a trovare le risorse per rendere permanente questa iniziativa.

Per quanto riguarda i Paesi in via di sviluppo, vengono ripristinati i contributi dell'Italia agli organismi internazionali, saldando il debito del Governo di destra, che al riguardo era inadempiente. Credo si tratti Credo si tratti di una iniziativa importante, perché riporta il nostro Paese all'interno del quadro internazionale, con una credibilità maggiore, e prevede 130 milioni per il versamento di una ulteriore quota, oltre a quella già destinata con il decreto di luglio, del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria.

vale a dire 2.225 milioni di euro. Si tratta di interventi rilevanti anche per la ricaduta ambientale in termini di abbattimento di CO2 nelle città in particolare:

una iniziativa importante per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina, sul trasferimento modale da e per la Sicilia per 75 milioni di euro;

al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici devono essere accompagnati da una certificazione relativa alla riduzione delle emissioni di gas serra. Si tratta di

Mi risulta che l'opposizione abbia presentato in Aula 449 emendamenti, un numero maggiore di quelli presentati in Commissione.

siamo perfettamente consapevoli della difficoltà di presentare a quest'Aula una questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 93 del nostro Regolamento, anche perché, nella sostanza, per quanto attiene ai riferimenti che farò alla legge di contabilità, l'avevamo già presentata e discussa in occasione

il Governo non si è fermato a un "tesoretto 1" e ha preparato un secondo decreto, cosiddetto tesoretto 2, quasi a significare una vendetta nei confronti del contribuente, del contribuente, che si prepara a sperperare ancora una volta quelle sostanze, quelle risorse, quelle rinvenienze al al Tesoro dello Stato che vengono dai sacrifici dei cittadini, perché è un cittadino cui il Governo continua a mettere le mani in tasca. Siamo contrari a che contrari a che il Senato continui a discutere di questo provvedimento. Siamo contrari, lo abbiamo detto in Commissione e vogliamo ribadirlo anche in questa sede, perché il provvedimento, così come quello precedente, è contrario alla legge di contabilità. lo voglio ricordare ai disattenti colleghi della maggioranza, ai colleghi che si disperdono nei meandri del palazzo e anche nel meandro del percorso

a fare. Siamo contrari, dicevo, con riferimento alla legge di contabilità, una legge rafforzata, discendente direttamente dall'articolo 81 della Costituzione, che non può essere variata con la legge di bilancio,

interesse, quella sbandierata attenzione che il Governo dice di avere per il Mezzogiorno giustappunto è provato con la sottrazione al Fondo per le aree sottoutilizzate di 1.100 milioni di euro. Come lo fa, signor Presidente? Con una copertura che trova fondamento nell'articolo 1 del decreto-legge: è stato fissato un indebitamento; l'indebitamento era il 2,9 per cento; le cose vanno meglio;

prevista in ogni finanziaria - di utilizzare migliori rinvenienze (cosa dice sempre quell'articolo 1?) per tre motivi, cioè

A questo punto cosa succede? Accade che gli obiettivi di indebitamento non sono quelli che erano stati fissati con i documenti legittimi stabiliti dalla legge di contabilità, la legge finanziaria, ma sono stati variati con un documento, il Documento di programmazione economico-finanziaria. Questo introduce un primo *vulnus*, cioè la possibilità che in corso d'anno un Governo,

motivo numero due: non sappiamo se le maggiori entrate sono permanenti, se sono strutturali, se sono delle entrate robuste. Il famoso documento che era previsto dal comma 4 della finanziaria da doversi produrre entro il 30 settembre non è stato prodotto e quindi ci ritroviamo nella impossibilità di vedere la loro strutturalità e la loro permanenza e quindi nella impossibilità di valutare se questo è in rispetto alla legge di contabilità o meno. Le maggiori entrate che vengono ad essere utilizzate non rispondono alla necessità terza del comma 4 dell'articolo 1 della finanziaria, ossia che queste vengano utilizzate ai fini ai fini degli obiettivi di cui al punto 3, e quindi equità fiscale, redistribuzione del reddito, interventi per lo sviluppo, perché come sappiamo benissimo

corrente e non c'è alcuna misura per quanto attiene alla fiscalità. A questo punto è logico ed evidente che stiamo realizzando un provvedimento che non è anticiclico ma è prociclico, ragion per cui speriamo tanto di non doverlo discutere e chiediamo all'Aula

anche perché un'ora fa la Commissione affari costituzionali ha licenziato un parere condiviso,

con la quale la Corte ha individuato, non solo la propria potestà di censurare i decreti-legge per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, ma anche degli

Tra questi elementi c'è, per esempio, la mancata adesione del contenuto delle norme del decreto-legge al preambolo del decreto stesso. Il preambolo di questo decreto-legge stabilisce che le ragioni di urgenza riposano nell'avvio di un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture e di investimenti. Ebbene, chiunque abbia avuto occasione di sfogliare il decreto‑legge sa che solo una piccola parte delle norme che lo costituiscono

È chiaro che questo rappresenta un *vulnus* non emendabile e su questo *vulnus*, anche se con caratteri non di perentorietà quali quelli che sto indicando, si è pronunciata la Commissione affari costituzionali. Un altro dato è quello della disomogeneità del provvedimento, perché esso contiene norme che vanno su vari capitoli, da quelli indicati, incapienti e infrastrutture,

al Governo e al relatore perché si facciano carico di una precisazione - che il commissario *ad acta* possa essere destinatario

Non vi è alcun motivo per giustificare un «trattamento di favore» del genere perché, o lo svantaggio è *in re ipsa*, oppure questo non può certamente dipendere solo dal fatto che le zone siano situate in località di

lotta all'evasione. Tuttavia, non abbiamo avuto il piacere di avere a disposizione la relazione al Parlamento, che avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 settembre scorso, sui risultati della lotta all'evasione, giunta

Signor Presidente, innanzitutto vorrei comunicare a tutta l'Aula - come ha già fatto il presidente Morando questa mattina

dall'opposizione e prevista dalla legge non sarà a conoscenza dell'intera Commissione; ciò al fine di garantire

nei nostri lavori. Anzi, l'augurio che esprimo a nome del Gruppo è che questo provvedimento possa essere approvato secondo il calendario stabilito dalla Presidenza.

Si tratta quindi dello stanziamento di fondi nel rispetto di un accordo siglato nel febbraio del 2007, che concerne il rinnovo di un contratto ormai scaduto.

per il Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria. Voglio ricordare come il nostro Paese si sia trovato nell'impossibilità di onorare impegni assunti anche dal Governo precedente, causa l'andamento della finanza pubblica. Mi sembra una misura su cui tutti si possa concordare della necessaria urgenza di riempire questo vuoto e di essere perciò coerenti rispetto agli impegni assunti a livello internazionale. Per non parlare poi dell'emergenza casa; come ci ricorda l'articolo 21, esiste un programma di edilizia residenziale pubblica che va anche a rispondere, il prima possibile,

alla data del 31 dicembre 2006 con scadenza alla fine di quest'anno. Così come l'articolo 32 risponde anche ad un giudizio della corte d'appello di Roma che ha concesso un rinvio della transazione tra ENEA e Finmeccanica che scade a dicembre del 2007; occorre pertanto intervenire con tempestività ed urgenza. L'articolo 33 disposizioni a favore dei soggetti talassemici: è un argomento delicato che coglie la sensibilità di noi tutti. Mi sembra davvero una corsa contro il tempo,

ricordando come la stessa misura prevista dall'articolo 44, la misura fiscale a favore dei cosiddetti soggetti incapienti, abbia una sua urgenza abbia una sua urgenza sociale, una situazione che risponde ad una marginalità sociale diffusa, ad una povertà certificata nelle sue dimensioni allarmanti anche dall'ISTAT:

che non sono, a mio avviso, meritevoli di essere accolte dall'Aula.

Discutiamo oggi di eventuali profili di incostituzionalità, ma non del particolare e specifico profilo della mancanza di presupposti perché, secondo il nostro Regolamento, questo profilo trova un momento trova un momento specifico di attenzione e di discussione che avrebbe dovuto essere, laddove i colleghi dell'opposizione avessero voluto, la richiesta di riportare in Aula il voto espresso dalla Commissione affari costituzionali sul punto. Poiché ciò non è stato fatto, ritengo corretto che in questo momento non si ritorni sulla questione;

Non mi pare poi che si debba andare molto oltre sul fatto che non sia opportuno procedere nell'esame del merito del decreto; mi riferisco alla questione Ho notato che il collega Ferrara ha voluto ricordare ancora una volta che questo decreto è servito e serve, nella sua opinione, a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. cittadini. Rispondo soltanto che la vera questione è da quali tasche vengano presi i quattrini e in quali tasche vadano a finire; ad esempio, dalle tasche degli evasori e vadano a finire nelle tasche delle fasce deboli della popolazione. Non arrivo a dire, con uno dei Ministri del mio Governo, che le tasse sono bellissime; francamente,

Senza le tasse non esisterebbe lo stato moderno e non esisterebbero i parlamenti, che sono nati appunto per decidere chi, come e quando fosse chiamato a pagare le tasse. Forse i colleghi dell'opposizione non sono consapevoli di essere portatori di questo peccato originale, di questa tara genetica; se l'onorevole Berlusconi ne fosse consapevole, dovrebbe forse dimettersi per coerenza da qualsivoglia carica pubblica.

possibile mancanza della necessità e dell'urgenza. La Corte, cioè, non censura l'eterogeneità del contenuto come tale, ma la censura in quanto quel pezzo in sé è mancante di necessità e di urgenza.

non avrebbe fatto questo richiamo se non fosse stato possibile che la questione fosse necessaria ed urgente a prescindere dal legame concettuale con il titolo.

quale bisogno avrebbe avuto la Corte di affermare nel caso in modo specifico quella mancanza di necessità e di urgenza? Non è quindi conclusivo l'argomento del collega Pastore. siano invece rilevanti le considerazioni da lui svolte per quanto riguarda alcune specifiche disposizioni. In particolare, voglio far riferimento agli articoli 4 e 35, che pure sono stati richiamati, e che toccano alcune delicate e complesse questioni. Nel primo articolo abbiamo una fattispecie di commissariamento. Cioè, nell'ambito della questione sanità, che tanto ci ha affaticato in relazione alla necessità di mettere sotto controllo la spesa sanitaria, si prevede la definizione di una procedura nella quale, ad un certo punto, di fronte all'inerzia della Regione interessata,

suscettibile di essere portata a comprendere addirittura l'adozione di atti normativi di rango primario: il commissario che fa le leggi.

Quindi, laddove prevediamo la possibilità di un commissario che assume atti a contenuto di generalità e astrattezza, dobbiamo pur sempre ritenere che siano atti che rimangono nell'ambito degli atti di natura amministrativa, mai degli atti di natura legislativa, né regolamentare.

e testuale formulazione, non impone una lettura diversa. Dunque, questa è la corretta lettura. Infatti, credo che la Commissione abbia espresso un giusto parere, nel senso della

deve intendersi nel senso che, laddove la contiguità sia di per sé produttiva di uno svantaggio, perché tale tale da creare condizioni comparativamente peggiori per un territorio rispetto ad altri (per esempio, a causa del minore costo di beni o servizi nel nel territorio della Regione limitrofa), in quel caso vi potrebbe essere un intervento di sostegno. Quindi, ci deve essere un'oggettiva e comprovabile diversità, non essendo la contiguità come tale suscettibile da essere assunta a fondamento di un vantaggio per questo o quel territorio. Anche in questo caso una lettura *secundum* *constitutionem,* che la norma nella sua formulazione testuale consente,

Presidente, ancora una volta, assistiamo nell'Aula del Senato ad un ostruzionismo da parte della maggioranza. Non mi scandalizzo certamente per questo e e nemmeno mi scandalizzo se fuori da quest'Aula c'è qualcuno che dà dell'analfabeta del diritto a qualcun altro. Non mi permetto di dare voti a nessuno né sul diritto né su altre materie, ma una cosa è certa:

ai voleri di pochi senatori che discutono, fuori da quest'Aula, le sorti del Governo. E noi siamo qui ad aspettare la fine della riunione del Consiglio dei ministri: l'Aula del Senato

Ripeto: non è possibile aspettare qui che si decidano le sorti di un Governo, e quindi le sorti di quest'Aula, fuori dall'Aula stessa. Coloro che sono fuori a discutere devono venire in Aula, chiedere la parola, intervenire e dichiarare cosa vogliano, così l'Aula avrà la possibilità di esprimersi. In questo momento, invece, c'è una mancanza di rispetto delle istituzioni che non ha precedenti nella storia della Repubblica italiana.

si difendano in molti modi. Uno di questi può essere quello di onorare i lavori parlamentari, come si sta facendo con gli interventi dei rappresentanti della maggioranza sulle questioni pregiudiziali. Un altro modo, che trovo assai meno consono alla tutela di quegli obiettivi, è per esempio il fatto di trasformare l'Aula del Senato in un luogo in cui, come spesso è accaduto in questi mesi, anche più volte sullo stesso argomento, si discute esclusivamente di mozioni, ferma restando ovviamente la tutela della libertà delle opposizioni di proporre atti di controllo o di impegno del Senato su molte questioni.

ha esitato il punto all'ordine del giorno che poteva riguardare, in qualche modo la soddisfazione di alcuni senatori della maggioranza e l'equivoco politico, la questione politica è stata ampiamente risolta. Si trovano tracce non abbondanti, presidente Matteoli, abbondantissime, nelle storie di tutti i Governi e anche di quello che ha preceduto l'Esecutivo in carica, di episodi di ostruzionismo della maggioranza, ma di quelli veri. Ne ricordo più di uno nel corso della passata legislatura, sancito non una questione puntuale, ma piuttosto un'aperta divaricazione di punti di vista all'interno della maggioranza, per esempio a proposito della

si svolga e che il Senato tranquillamente voti. Non c'è da parte della maggioranza neanche un attimo di esitazione strumentale rispetto a questo. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, mi limiterò a replicare puntualmente alle questioni di sostanza sollevate

del 2006 che disciplina le regole alle quali si dovrebbe ispirare la manovra di finanza pubblica per il 2007. Nella questione sospensiva presentata si fa però riferimento solo alla prima parte del comma 4.

poiché il comma 4 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che dovrebbe essere, appunto, una norma di riferimento per i nostri comportamenti tecnici, ci impone di fare esattamente quello che è scritto nel decreto-legge n. 159 in esame. Lo voglio ricordare, perché è scritto

a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse». Il decreto-legge n. 159, signor Presidente, onorevoli colleghi, fa esattamente questo. Ha preso atto, con riferimento alle disposizioni di assestamento, che vi è stata un'entrata maggiore e permanente, ormai stabilizzata, dovuta, appunto, alla lotta all'evasione fiscale, comunque alle maggiori entrate ha destinato una prima parte - lo dice il decreto-legge stesso - a quegli obiettivi di finanza pubblica che sono stati ritenuti urgenti e una parte successiva, con gli articoli da 2 in poi, ad una manovra di equità fiscale fiscale e sociale, dando rimborsi a coloro che non hanno potuto presentare nemmeno una dichiarazione dei redditi, dando sostegno ai lavoratori socialmente utili e dando supporto alle categorie svantaggiate. Se dovessimo

Qualsiasi altro strumento avrebbe potuto richiedere una legislazione di natura differente, ma in Commissione abbiamo svolto un'analisi molto puntuale di ciascuna delle disposizioni e mi sento di poter dire che non ve n'è nemmeno una che non svolga i suoi effetti nella immediatezza o perché attraverso caratteri di natura procedimentale pone le condizioni per attività che devono essere svolte successivamente o addirittura perché gli stessi effetti ed esiti economici e finanziari si sviluppano nell'ambito degli stessi sessanta giorni di vigenza del decreto. Ha ragione il collega Pastore quando dice che, sulla base di una ormai nota sentenza della Corte costituzionale, il Governo avrebbe dovuto essere meno laconico nel titolo e nel preambolo. Anche noi abbiamo fatto questa osservazione, l'abbiamo condivisa, ma è un auspicio che non possiamo che riferire alla decretazione successiva. Peraltro, voglio ricordare che, se per il preambolo non vi sono strumenti, per il titolo la stessa Aula potrebbe adottare degli accorgimenti che alla fine comprendano tutti i punti, anche se, signor Presidente, onorevoli colleghi, devo riconoscere che nella laconicità il titolo fa però riferimento a "interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale". E credo che tutte le disposizioni (che riguardano finanza pubblica, interventi infrastrutturali e recupero di soggetti che si trovano in condizioni di svantaggio) possano essere racchiuse in questo titolo, anche se assai laconico. Sono state poste, signor Presidente, onorevoli colleghi, anche alcune questioni che fanno più riferimento all'incidenza nel merito. Per quanto riguarda l'articolo 4, sul quale è stata sollevata una questione che concerne la scelta del commissariamento *ad acta* per provvedimenti di natura normativa, ordinamentale, gestionale e amministrativa delle Regioni, si è voluto fare un approfondimento di carattere tecnico. Ci rendiamo conto e non possiamo non prendere atto del fatto che si tratta di materia concertativa, che le disposizioni dell'articolo 4 sono il frutto della Conferenza Stato-Regioni, che si tratta di atti sostanzialmente concordati, che i piani di rientro sanitari fanno parte appunto di quell'accordo che lo Stato e le Regioni hanno raggiunto nel momento in cui la manovra di finanza pubblica concernente la spesa sanitaria è stata concordata le stesse Regioni hanno riconosciuto tali atti come strumenti procedurali idonei. Abbiamo ritenuto, però, di dover andare oltre quello che lo stesso Stato e le stesse Regioni hanno concordato: abbiamo riconosciuto il valore di carattere generale della disposizione della legge La Loggia, proprio in relazione alla sua capacità di dare attuazione all'articolo 120 della Costituzione abbiamo richiamato il Governo - così come richiamiamo l'Aula - a verificare se le disposizioni procedimentali concernenti il commissariamento *ad acta* siano coerenti con quelle previste dalla normativa di carattere generale della legge La Loggia, che abbiamo voluto citare nel nostro parere. Abbiamo anche richiamato, signor Presidente, il rispetto dell'articolo 120 della Costituzione. L'ha detto molto bene il collega Villone: la legge La Loggia è meramente attuativa e la Costituzione non va richiamata ogni volta perché vige, al di là dei nostri richiami, nelle leggi attuative. Di fatto, però, abbiamo voluto precisare che questo commissario *ad acta*, nel momento in cui potrà - perché potrà compiere anche atti normativi nell'adempimento dei propri doveri (concernenti appunto l'attuazione dei piani di rientro che le Regioni non avranno attuato), Regioni non avranno attuato), certamente non potrà compiere atti di legislazione generale; non potrà nemmeno compiere atti di normazione di carattere primario che non abbiano esplicito, espresso e vincolante riferimento proprio a quel commissariamento per quei piani di rientro sanitario che gli sono stati affidati in sostituzione appunto di una Regione che non vi ha adempiuto. Infine, signor Presidente, i colleghi Villone e Pastore hanno posto una questione che credo rilevante, relativa alle zone di confine, principio che per la introduciamo nel nostro Paese tra Regione e Regione e non fra Stato e Stato. È chiaro che questo va vincolato ad una situazione di effettivo svantaggio, che deriva dalla posizione limitrofa rispetto a queste Regioni. Penso che che possiamo concludere che il lavoro che abbiamo svolto in Commissione e che il collega Pastore ha voluto citare ci possa tranquillizzare. Le ragioni che ho espresso sulla sospensiva e quelle che abbiamo convenuto in Commissione affari costituzionali sulle pregiudiziali ci possono indurre tranquillamente a respingere tali questioni.

rispondono ad emergenze alle quali è necessario dare una risposta. Se mi permette, credo di essere finito in quest'Aula per puro caso, non sono un esperto di diritto costituzionale,

e da uomo del popolo (perché, come si dice dalle mie parti, ho fatto la terza media in bicicletta perché a 15 anni sono dovuto andare a lavorare...

I problemi che sono stati sollevati, come ha detto anche il collega Sinisi, sono stati raccolti e alcuni punti critici sollecitati sono stati portati all'attenzione dell'Assemblea, ma nel complesso non c'è stata proprio una

esiste davvero nel nostro Paese una emergenza sociale di cui anche noi, anche noi, anche la maggioranza, parla, quando affronta i dibattiti sulla questione della perdita del potere di acquisto. Esiste una questione grande come una casa che

questo. Sarebbe più utile, forse, anche se diventa più complicato svolgere un dibattito pubblico, discutere nel merito: allora, se l'opposizione non è d'accordo su alcuni provvedimenti di carattere sociale lo dica chiaramente, senza porre il problema della pregiudiziale di costituzionalità.

vere: conveniamo sempre tutti che soprattutto il trasporto pubblico locale sia non solo carente ma versi in condizioni inaccettabili per i passeggeri.

Colleghi, c'è una richiesta del senatore Calderoli ai termini dell'articolo 98

Presidente, non so se, dopo che la Commissione bilancio ha esaminato

il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è già stato ascoltato. Quindi, chiedo alla Presidenza di valutare l'ammissibilità di questa richiesta.

che finalmente oggi sono tutti presenti, perché non è capitato di sovente, quindi ci hanno provato seriamente a dare la spallata;

al CNEL, è esattamente quella che è già stata proposta dal senatore Boccia, che però voglio, se lei me lo consente per pochi secondi, arricchire. Faccio notare ai colleghi, in particolare al senatore Calderoli, che non ci troviamo in presenza di un qualsiasi decreto. Tanto è così, che noi abbiamo deciso in Commissione bilancio, con parere assolutamente condiviso, che la discussione generale su questo decreto fosse unita a quella sulla finanziaria e a quella sul bilancio, dimostrando così che è comunemente accettato che tale provvedimento sia parte organica della manovra di bilancio e quindi della sessione di bilancio. Così è al punto che, durante le audizioni, moltissimi auditi si sono pronunciati e hanno formulato pareri - penso, ad esempio, all'ISTAT prevalentemente sulle misure contenute nel decreto-legge (mi riferisco, per esempio, alla misura contenuta nel provvedimento a proposito degli incapienti), dando valutazioni sugli effetti della misura del provvedimento sulla manovra nel suo complesso.

che lei, signor Presidente, ha autorizzato, perché non avremmo mai potuto tenere l'incontro con il CNEL se lei non lo avesse autorizzato. Per queste ragioni, a mio avviso, la richiesta del senatore Calderoli è del tutto inammissibile. Presidente, voglio solo ricordarle che lei aveva già chiamato la votazione. È sempre un piacere ascoltare il senatore Boccia, ma lei aveva già chiamato la votazione. Lei, Presidente, ha detto: "È aperta la votazione"; dai banchi della maggioranza)* dopodiché ha dato la parola al senatore Boccia, ma vedo difficile che lei possa tornare indietro, perché le argomentazioni del senatore Boccia non credo siano sufficienti. Ha detto che noi facciamo ostruzionismo; va bene, vuol dire che facciamo ostruzionismo come avete fatto voi fino a pochi minuti fa, ma non mi sembrano questi argomenti sufficienti per farle cambiare idea. Quindi, la invito a mettere in votazione la richiesta del collega Calderoli.

dopo il rigetto della pregiudiziale e della sospensiva, una posizione politica di rilievo, per cui, in tranquillità, posso dire che, essendo stato ascoltato con il mio permesso, credo se ne possa fare a meno; questa è la mia decisione. La Commissione lo ha ascoltato. Come voi sapete, io riconosco l'autorevolezza del senatore Morando, ma quando non sono d'accordo glielo dico, come è accaduto in altre occasioni in Assemblea. Questa volta mi pare assolutamente convincente, tratta di un parere che può essere chiesto anche in due giorni, ma che non tocca il merito e le posizioni politiche in questa discussione. Pertanto, mi sento, in tutta tranquillità, di dire che il CNEL è già stato ascoltato. Quindi, ritengo questa proposta non ammissibile.

Quello che viene riferito nel corso delle audizioni non costituisce atti ufficiali: vengono alcuni rappresentanti del CNEL, ma non vi è un pronunciamento del CNEL,

non è stato dato perché non credo che si possa dire che quest'Aula ha il parere dell'ISTAT, ancorché audito in Commissione. Il Regolamento prevede questo, il limite è posto dalla materia

parlamentare, copia della relazione al Parlamento del Ministero dell'economia e delle finanze sui «Risultati della lotta all'evasione», inviata dal ministro Tommaso Padoa-Schioppa. La presente relazione è stata redatta dal vice ministro, onorevole professor Vincenzo Visco, nell'ambito delle deleghe a lui intestate. La data è

Questo argomento era parte fondamentale della questione pregiudiziale che avevamo posto, perché ci apprestiamo a discutere della conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre che disperde 7,6 miliardi di euro sulla base del presupposto che sono improvvisamente emerse quest'anno maggiori entrate, che queste maggiori entrate sono frutto della lotta all'evasione e che esse sono strutturali e permanenti. Senza questi elementi, il decreto che il Senato andrà a convertire in legge è privo di ogni base giuridica di riferimento. A questo punto, signor Presidente, vorrei che lei verificasse quando

del Regolamento. Ciò risolve il problema relativo al parere reso in Commissione, atteso che esso possa e debba essere recepito non soltanto dai componenti della Commissione - che sono deputati ai più stretti lavori inerenti alla formazione delle leggi con finalità di politica economica, sociale (ragione per cui un senatore esterno alla Commissione deve essere messo nelle condizioni, non già per specifica volontà, per atto di predisposizione

sono stati ricevuti ed elaborati dall'Aula, ragion per cui le prerogative che discendono al parlamentare dall'articolo 98 possono essere salvaguardate soltanto da un voto dell'Assemblea. Questo è il motivo per cui non esistono precedenti, così come richiamato dal senatore Calderoli e il fatto che lei voglia decidere in modo diverso costituisce - se mi permette, con il dovuto rispetto - un *vulnus* notevole per i lavori e per la formazione delle leggi con rilevanza economica, sociale e di programmazione economica.

al procedimento legislativo, l'aver acquisito il parere esplicito e formale del CNEL sul decreto‑legge al nostro esame, mi pare che chiuda oggi la questione.

Presidente, lei ovviamente farà quello che vuole e mi pare che questa discussione si sia anche svuotata di senso politico

tanto che ha concluso, dopo una brevissima consultazione con quelli che lei chiama i suoi collaboratori, annunciando all'Aula il passaggio al voto. Ora, io non capisco il motivo per il quale non si voglia procedere a questo atto dovuto, atteso che non mi sembra esistano elementi di pericolosità

perché in questo modo si produce un'incertezza nell'Aula. Noi abbiamo una visione tale delle decisioni della Presidenza per cui non è possibile che ad ogni stormir di fronda si possa cambiare opinione, atteso che qui non c'è opinione da cambiare, ma solamente la necessità di esprimersi con un voto, così come è stato richiesto. Presidente, valuti con attenzione tutto questo perché anche quello che lei ci ha detto, pensando di correggere la sua decisione, in effetti l'ha rafforzata.

Non si faccia richiamare dalle sirene della maggioranza; credo che si debba far chiamare di più dalla sua coerenza che spesso, in modo chiaro e determinato, ha dimostrato a quest'Aula. Non succede nulla per un voto!

Senatore, confermo la necessità di portare quest'argomento alla Giunta per il Regolamento, Voglio soltanto sottolineare che

Al secondo comma dell'articolo 98 del nostro Regolamento, infatti, si dice espressamente che il parere viene pubblicato, subito dopo la trasmissione, in un apposito stampato allegato al disegno di legge. È evidente *ictu* *oculi* a tutti i senatori che al disegno di legge non è stato allegato alcun apposito stampato recante il predetto parere

specifico procedimento attraverso cui l'Assemblea richiede un parere al CNEL, ma non prende atto di una decisione autonoma del CNEL attraverso cui formula il parere. Possiamo aggiungere un'ulteriore considerazione. Nel formulare la richiesta al CNEL, l'Assemblea può chiedere specifici elementi di parere, che il CNEL, nella sua autonoma iniziativa, adottata in questa occasione, non poteva conoscere.

che l'Assemblea e le Commissioni possano chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi e indagini previa definizione dell'oggetto e della finalità; i risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL. Siamo pertanto nella fattispecie di una richiesta

della legge finanziaria dello scorso anno, come sarebbe stato necessario in ottemperanza ad una richiesta esplicita del Parlamento. Inoltre, questa relazione fa filosofia sulla politica tributaria, ma non fornisce i risultati della lotta all'evasione, come invece il Parlamento aveva chiesto. Detto questo, signor Presidente, c'è un'altra questione sulla quale vorrei richiamare la sua attenzione.

per 40 miliardi di euro, rispetto alla quale il Parlamento è estraneo in tutto il processo di definizione. Questa è una materia che non può essere contenuta nel decreto-legge se vogliamo un ordinato svolgimento dei nostri lavori. Presidente, richiamo la

Signor Presidente, onorevoli colleghi, e soprattutto onorevoli colleghi della maggioranza (e non perché non mi voglia rivolgere ai colleghi dell'opposizione), ai colleghi dell'opposizione), bisogna riconoscere che il confronto in atto al Senato sul decreto fiscale si svolge in un clima tutt'altro che sereno per il Governo. La coalizione di centro-sinistra appare un convoglio i cui passeggeri non sono affatto d'accordo sulla destinazione. Esiste una fibrillazione politica che si accompagna ad un vasto e diffuso disagio sociale, che rischia di far velo ai numerosi e positivi provvedimenti che il Governo ha varato (e il decreto al nostro esame è uno di questi). Il risanamento economico e finanziario non è qualcosa di estraneo alla soluzione dei problemi sociali drammaticamente aperti nel nostro Paese. Senza una crescita economica superiore a quanto previsto all'inizio della sessione di bilancio dell'anno scorso e senza un'importante emersione di parte dell'evasione fiscale non saremmo qui a discutere di come usare le risorse in più rispetto alle previsioni. È importante che il Governo rivendichi a sé i meriti di questa condotta ed è altrettanto importante che non abbandoni la strada del rigore. Vi sono tuttavia in questo decreto, onorevoli colleghi, alcuni punti critici e ad e ad alcuni di essi, come senatori della Costituente socialista, abbiamo cercato di porre rimedio con pochi e mirati emendamenti. L'anno scorso si è deciso che tenendo presenti le condizioni politiche e sociali del nostro Paese le risorse recuperate con la lotta all'evasione fiscale sarebbero state prioritariamente destinate ad interventi di sostegno ai cittadini e alle cittadine più povere e in difficoltà, utilizzando anche la leva fiscale, poiché è notorio a tutti che la pressione fiscale nel nostro Paese è troppo alta.

Per questo non siamo contrari alla presenza nel decreto di importanti spese in conto capitale, dalle infrastrutture all'edilizia residenziale pubblica; anzi, ci rallegriamo che gli investimenti pubblici rispetto alle spese correnti aumentino anche con la prossima legge finanziaria. o almeno riqualificare la spesa corrente e aumentare la spesa in conto capitale dovrebbe essere una linea guida essenziale in un Paese come il nostro, dove mancano infrastrutture e ricerca. In questa direzione la riduzione del debito pubblico, la qualificazione della spesa, le misure per una maggiore equità sociale sono una priorità. Ci chiediamo su questo fronte se proprio non si poteva fare di più. Certo che si poteva fare di più. Per esempio, la misura proposta inizialmente dal Governo in favore degli incapienti, diciamolo, non ci ha convinti in pieno. Quello che non ci è piaciuto delle misure proposte per la parte più indigente della nostra società è principalmente il fatto che di fronte ad una grossa spesa per lo Stato - quasi 2 miliardi di euro - la sua suddivisione tra un gran numero di persone implicherà un beneficio per ogni cittadino alquanto limitato, per di più temporaneo. Il carattere *una tantum* della misura è appunto il secondo aspetto che non ci convince. Si dirà che non possiamo sapere se l'extragettito ha natura strutturale e dunque le risorse disponibili erano esse stesse *una tantum*; è vero, ma è per questo che sarebbe stato opportuno dedicarla agli investimenti che favorissero i più poveri e gli emarginati da un punto di vista strutturale. Per esempio, è per questo che le nuove risorse dedicate all'edilizia residenziale pubblica sono la misura sociale che più ci convince. Con il primo emendamento che abbiamo presentato, abbiamo cercato di migliorare, e non eliminare, la misura in favore degli incapienti, degli incapienti, innanzitutto puntando a qualificare meglio la platea dei beneficiari, per evitare il ridicolo di rischiare di dare soldi agli evasori. Il vantaggio deve andare a chi è assistito dai servizi di assistenza sociale dei Comuni, a nostro giudizio, a chi è disoccupato, a chi è lavoratore dipendente, ai pensionati tra i più poveri; quindi, avere come riferimento le condizioni economiche familiari e non già il reddito individuale. Il nostro obiettivo è che la riduzione del numero dei destinatari e la selezione di quelli che versano in maggiore difficoltà possano portare ad un aumento del beneficio spettante ad ognuno, con un ancora più visibile miglioramento delle condizioni di vita, rispetto a quanto ipotizzato inizialmente dal Governo. Inoltre, questa migliore selezione dei beneficiari dovrebbe portare, secondo i nostri calcoli, ad una riduzione della spesa per lo Stato. Abbiamo dimostrato che è possibile trovare almeno 200 milioni di euro per l'assistenza all'infanzia. Il convergente lavoro nell'ambito della maggioranza ed il sostanziale accoglimento di alcune delle nostre proposte ci hanno consentito pertanto di ritirare l'emendamento di cui parlavo. L'extragettito di cui discutiamo dimostra come la qualità della spesa a sostegno dell'occupazione, lo sviluppo e la crescita economica siano la maniera migliore di risanare i conti pubblici. L'altra maniera - non c'è dubbio alcuno - è il recupero dell'evasione fiscale. Tale risultato può e deve essere ottenuto con l'individuazione e la sanzione degli evasori, ma anche stabilendo un rapporto corretto tra Stato e cittadino. È per questo che ci sembra ben strano, in un momento in cui agli italiani chiediamo di fare sacrifici per risanare i conti e ridurre il debito, che tante importanti risorse - e ce ne sono tante, onorevoli colleghi - vengano sprecate, disperse in mille rivoli e in autentiche regalie. E non stiamo parlando di cittadini indigenti. C'è un nostro emendamento al decreto, che manteniamo, che si riferisce all'8 per mille, in cui proponiamo, senza enfasi laiciste, una riflessione. Secondo le stime del Governo, solo il 41 per cento dei contribuenti destina il proprio 8 per mille a qualcuna delle opzioni proposte. Di questi, la maggioranza sceglie la Chiesa cattolica. Come ben sapete, lo Stato decide di destinare invece quasi tutte le risorse dell'8 per mille sulla base dell'indicazione di una minoranza dei contribuenti, ovvero destina l'inoptato ad un'ulteriore redistribuzione, pari percentualmente alle opzioni dichiarate, con il risultato di assegnare la quasi totalità delle risorse alla Chiesa cattolica. Insomma, chiediamo ai contribuenti di pagare le imposte e poi assegniamo risorse senza il consenso degli stessi e senza che neppure lo sappiano. Noi, sia chiaro, onorevole Presidente, non intendiamo fare battaglie ideologiche contro la Chiesa, che svolge meritoriamente, con altre confessioni religiose o associazioni laiche, compiti di assistenza sociale e non proponiamo l'abolizione dell'8 per mille. L'assegnazione delle risorse, però, deve avvenire sulla base di scelte consapevoli e nell'assoluto rispetto del principio della libera manifestazione di volontà del contribuente, che invece nel nostro caso viene aggirata, per non dire - peggio - raggirata. perciò di destinare l'8 per mille che non viene destinato dai cittadini a nessuna opzione al proseguimento, anche nel 2008, del piano straordinario di edilizia residenziale, avviato con questo decreto. Si tratta di mezzo miliardo di euro: davvero un aiuto concreto a tante persone in condizioni di disagio.

La nostra iniziativa è tesa ad ottenere un'azione di Governo più incisiva ed efficace. Non chiudiamo certo gli occhi di fronte alle gravi contraddizioni che pervadono la maggioranza e il Governo. Siamo convinti che, una volta varata la manovra economica, bisognerà arrivare ad un chiarimento politico e strategico. Occorrono un nuovo programma Certo, così non si può andare avanti. Continuiamo a pensare che, con la nascita del Partito Democratico, bisogna ancora dimostrare che si rafforza il Governo e che le giuste istanze e le rivendicazioni provenienti dalla manifestazione di sabato scorso meritano di ricevere risposte da un'iniziativa parlamentare e di Governo innovativa e perciò

*(AN)*. Signor Presidente, ovviamente debbo svolgere questo mio intervento in discussione generale avendo letto soltanto la metà del punto fondante del dibattito che stiamo svolgendo, cioè la relazione sui risultati della lotta all'evasione fiscale, atto dovuto da parte del Governo entro il 30 settembre 2007 pervenuto al Senato soltanto oggi pomeriggio. Ebbene, la prima riflessione che nasce dalla lettura di queste prime pagine è che questa sia una relazione clamorosa. Mi rendo conto che non interessa molto al Senato e ai colleghi senatori, anche perché credo che pochissimi tra i colleghi abbiano già a quest'ora a disposizione questa relazione, atto dovuto - ripeto - da parte del Governo entro il 30 settembre. avendo io tentato di leggerla (sono arrivato soltanto a pagina 6 di un documento di 33 pagine), mi rendo conto che neanche i colleghi hanno potuto prenderne visione. Signor visione. Signor Presidente, questa relazione è un fatto politico clamoroso. Il Governo ci viene a dire in quest'Aula che sono stati recuperati 23 miliardi di imposte evase, e ce lo dimostra sulla base di un'analisi dell'andamento del gettito nell'anno 2006. Ebbene, signor Presidente, questa è la controprova di quello che questo Governo ha commesso nel dicembre 2006, truccando i conti per l'anno 2007. Francamente avrei consigliato al Governo di scegliere un numero diverso e di non dire che il maggiore gettito ammonta a 23 miliardi di euro nel 2007;

nella quale il Governo afferma che già sulla base del consuntivo 2006 si poteva perfettamente calcolare che il gettito di quest'anno sarebbe arrivato a 726 miliardi e non a 703 miliardi, quelli iscritti in bilancio nel dicembre dello scorso anno.

Il Governo mette per iscritto e documenta che nell'anno 2007 ha scritto un numero falso in bilancio (703 e che con i dati disponibili per l'anno 2006 avrebbe potuto e dovuto scrivere 726 miliardi. Oggi ci mette una pezza

che questo effetto sia dovuto alla lotta all'evasione. E l'uso dell'espressione inglese *tax compliance* non inganna nessuno, perché indica semplicemente la buona volontà dei contribuenti. Magari fosse stata una maggiore buona volontà dei contribuenti. Con questo documento, che - ripeto - forse non a caso il Ministro dell'economia non ha firmato

Sarebbe opportuno che le alte magistrature contabili e le alte magistrature della Repubblica - spero ne abbiano il tempo - leggessero attentamente questo documento (la relazione inviata al Parlamento dal Ministero dell'economia e delle finanze sui risultati della lotta all'evasione), nello

in Commissione, il presidente Morando ha dovuto ulteriormente sollecitare il Governo a consegnare questa relazione (quindi, è falsa anche la data).

la decisione, una volta accertate la strutturalità e la permanenza del maggior gettito, di ridistribuirlo per fare equità sociale e sviluppo (l'ha ricordato oggi il relatore Ripamonti). questo è il secondo *boomerang*, perché il dettaglio delle voci di questo decreto dimostra che esso non ha niente a che vedere con lo sviluppo,

senza dare la concreta certezza che esistano anche per gli anni futuri e provengano dalla lotta all'evasione (non dall'aver commesso un falso in bilancio),

analizzano in modo preciso i dati del 2006, cioè quel consuntivo sulla base del quale il Governo doveva apporre numeri giusti nel bilancio del 2007. Occorre guardare i resoconti stenografici della Commissione e dell'Aula per ricordare che il Governo a dicembre rifiutò quello che scrive oggi,

che già allora avevano elementi di strutturalità. Quindi, deve rispondere alle alte magistrature della Repubblica e contabili di tale mancata registrazione di gettito. Mi avvio a concludere ricordando il terzo Anche qui, il dettaglio degli articoli e dei commi di questo decreto, raccolti in una piccola tabella, voce per voce, il cui totale arriva a 7,6 miliardi di euro, è disperso su circa 200 diversi provvedimenti, che oscillano singolarmente da un valore compreso tra 5 e 400 milioni,

ad una categoria di incapienti che probabilmente, proprio sulla base dei dati sull'evasione fiscale, rischiano di andare molto ad incapienti che risultano tali per evasione fiscale e magari

dobbiamo avere la consapevolezza di comunicare al Paese eventualmente anche una radicale differenza e difformità di valutazione sulle misure di politica economica fiscale e sociale che il Governo intende assumere e che il Senato si appresta a votare. Forse servirebbe a tutti (alla democrazia, al Paese, alle istituzioni)

con la situazione difficile in cui versano il Paese e l'economia dell'Occidente (italiana, europea e persino degli Stati Uniti d'America). Siamo in presenza di uno sconvolgimento degli equilibri mondiali. L'India e la Cina ormai rappresentano i fattori trainanti che da questo punto di vista determinano condizioni tali da incidere pesantemente sui rapporti di scambio, le divisioni del lavoro, la distribuzione delle risorse, il destino perfino del nostro Pianeta sono in grado di scaricare sull'Europa e - pensate un po' - anche sull'Italia, gli effetti sia dei fattori trainanti che dei rallentamenti. Basta vedere quali sono stati gli effetti sull'economia europea loans* degli Stati Uniti, per renderci conto di come nel Regno Unito è fallita una banca la Banca europea è stata costretta ad intervenire in maniera pesante, così come aveva fatto la *Federal Reserve* americana. Tutti noi sappiamo (di questo dovremmo occuparci) che coloro i quali, con prudenza e sacrifici, si sono caricati in questi anni e in questi mesi di un mutuo per comprare la casa, o altro bene a tasso variabile, nel corso di questo anno e mezzo si sono visti aumentare in maniera significativa la rata del mutuo, al punto tale che parecchi non ce la fanno e qualcuno, oltre a non farcela, non ce la fa più a resistere, a vivere e si uccide, se quello che abbiamo letto sulle cronache

decreto in esame, come l'insieme della manovra, che affronteremo anche con la finanziaria e l'ulteriore provvedimento sul *welfare*, non rappresenta la svolta epocale delle condizioni economiche e sociali, rappresenta una svolta rispetto all'anno scorso: mentre allora avevamo dovuto fronteggiare, in primo luogo, l'esigenza di coprire i *deficit* a livello interno ed internazionale, quest'anno si compie una operazione che non piace a tanti (non piace a molti editorialisti del «Corriere della Sera»; non piace da questo punto di vista neppure al Governatore della Banca d'Italia, se ne faccia una ragione perché non può pensare che sempre e comunque sono tutti ai suoi ordini; non va bene neppure al Presidente della Confindustria, anche lui se ne faccia una ragione): c'è qualcosa che va nella direzione della redistribuzione - guardate un po' - della spesa pubblica. Allora, quando la spesa pubblica è indirizzata a risolvere problemi che valgono 5 miliardi di euro in ragione del cuneo fiscale a beneficio delle imprese, tutto va bene; quando la spesa pubblica va in direzione di 1.900 milioni di euro per gli incapienti

componente della famiglia che non arriva ad un livello di reddito tale da dover pagare le tasse: immaginate la ricchezza, siamo al di sotto dei 7.550 euro l'anno e si dà un minimo di redistribuzione in questa direzione, a quel punto si levano gli alti lai: per carità, la spesa pubblica sta andando fuori controllo. Un'altra quota di spesa pubblica è orientata allo sviluppo, alle infrastrutture, alle Ferrovie, all'ANAS. C'è da ragionare molto su come

alle infrastrutture, fisiche e telematico-informatiche, per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno, piuttosto che - come appare ancora dalla distribuzione - alle Regioni del Centro-Nord, non per ragioni di campanilismo

terreno e quote di arricchimento indebito (quei 90 miliardi di euro di cui parlano i giornali oggi) e contemporaneamente si contribuisce alla crescita economica del Paese; nella misura in cui il Mezzogiorno contribuisce alla crescita è evidente che anche il Nord del Paese ne può trarre un grande beneficio. Di questo stiamo parlando, di questo - voglio

individua in questa manifestazione anche gli elementi di criticità, di ritardo. Noi siamo animati dall'ansia di fare di più e meglio in questa legislatura con questo Governo; pensiamo che ci siano elementi importanti che sono stati definiti, sia con il concorso del Governo, sia con la partecipazione attiva nella discussione in Commissione,

che in una legge di bilancio, in una legge dello Stato, si prevede un finanziamento per l'edilizia residenziale pubblica.

n. 9 del 2007, abbiamo 550 milioni di euro per la politica della casa; abbiamo un progetto per recuperare una parte del demanio militare da devolvere e orientare, sì ai servizi, ma anche all'abitazione; abbiamo un rilancio dei contratti di quartiere. Abbiamo lavorato

insieme alla manifestazione di sabato, rivendicazioni correnti e concrete. Continueremo a sviluppare questo ragionamento. Lo approfondiremo durante la discussione della finanziaria e anche successivamente. Siamo convinti, nel confronto interno alla maggioranza, ma anche nel confronto e nella capacità di far pesare il Paese sulle scelte del Governo, di poter ritrovare una sintonia forte

Signor Presidente, un attimo fa è stato detto che questa manovra non piace a tanti. Ci sarà pure un perché. Non piace - credo - alla stragrande maggioranza dei cittadini italiani per il fatto che non affronta organicamente tutti gli aspetti sociali. Non piace poi perché non persegue un percorso di risanamento finanziario e di riduzione del rapporto

non piace a tanti. Infatti in questo periodo le istituzioni economiche e finanziarie, nazionali e internazionali, esprimono tante critiche all'operato del Governo sulla manovra di finanza pubblica. Dopo il Fondo monetario internazionale,

di aver fatto troppo poco per il risanamento. Questo mi pare che sia un fatto fondamentale, perché se in una famiglia non c'è una situazione sana, il futuro

di utilizzare le entrate fiscali per ridurre il *deficit* e il debito. Credo che su tale aspetto e su tale affermazione non si possa che concordare. Al contrario, invece, la manovra non solo - come ho detto prima - non persegue il risanamento dei conti pubblici, ma non riduce e neppure riqualifica la spesa pubblica. Il commissario agli affari monetari ed economici Almunia accusa palesemente il Governo Prodi di utilizzare buona parte dell'extragettito per aumentare la spesa, in particolare con il decreto sul *welfare*. È un atteggiamento, a mio modo di vedere, colpevole ma sopratutto imprevidente, perché pone l'Italia in una condizione di ulteriore emergenza, anche per l'immediato futuro, proprio a causa dei livelli *record* della spesa e dei debiti dello Stato. Infatti, la manovra economica ha addirittura la stravaganza di accrescere il *deficit* pubblico rispetto all'andamento tendenziale senza l'intervento del Governo: invece dell'1,8 per cento si passerebbe al 2,2 Come ho detto, ci sono - e lo sappiamo - le condizioni per investire a favore del risanamento e quindi della capacità del nostro Paese di ridurre gli *handicap* di natura economica e finanziaria per essere un Paese più competitivo ed efficiente non soltanto in Europa, ma nel cosiddetto contesto internazionale globalizzato. Se non siamo nella condizione di poter essere competitivi e di mettere in atto tutte quelle per poterlo diventare, è chiaro che miniamo il nostro futuro in ragione della grande capacità e dell'aggressività non soltanto delle economie tradizionali ma anche dei Paesi emergenti; penso evidentemente alla Cina, all'India, ad alcuni Paesi dell'America latina. Allora veramente è colpevole da parte del Governo, a mio modo di vedere, non mettere in atto quelle misure che possono renderci più competitivi e creare anche quelle condizioni per per un migliore sviluppo economico e sociale; questo mi pare che sia il fatto fondamentale. Naturalmente, l'aumento della pressione fiscale colpirà le famiglie e le imprese, che in questo contesto internazionale - come dicevo poc'anzi - e anche con la moneta forte avranno ulteriori difficoltà non solo ad incrementare le proprie quote di mercato, ma addirittura a mantenere quelle attuali; e chi perde quote di mercato innesca un processo negativo per la stessa economia. Per quanto riguarda le imprese, a fronte delle aliquote IRES e IRAP, vi è l'ampliamento delle basi imponibili; vengono ridotte le aliquote, ma si ampliano le basi imponibili. La conseguenza potrebbe essere per le imprese una parità di saldo, ma per alcuni osservatori addirittura dovrebbe invece avvenire una crescita del prelievo fiscale. Quindi sono condizioni indubbiamente molto difficili. Voglio soffermarmi sull'IRES: l'aliquota scende dal 33 per cento al 27,5 per cento, ma l'ampliamento della base imponibile si realizza con un nuovo limite della deducibilità degli interessi passivi e con l'abolizione ad esempio degli ammortamenti anticipati.

di deduzione dal reddito degli ammortamenti anticipati e accelerati per i beni strumentali significa creare le condizioni negative per aziende in termini di possibilità di migliorare la capacità produttiva e soprattutto la capacità qualitativa dei nostri prodotti. Quindi, questo è un provvedimento che da una parte indebolisce l'intero settore dei beni strumentali del nostro Paese (un settore veramente fondamentale che - lo ricordo - nell'anno passato ha avuto un beneficio di 12,5 miliardi come bilancia dei pagamenti) e dall'altro il fatto di ridurre la possibilità di un ammodernamento delle tecnologie produttive innesca indubbiamente un processo di depressione della nostra industria, della nostra capacità di essere competitivi a livello mondiale. Questo provvedimento è estremamente

un esempio: lo sgravio ICI è parziale ed è *una tantum*. Gli sgravi, inoltre, saranno compensati dall'incremento del carico tributario

atteggiamento veramente incomprensibile, che non guarda al futuro e che anzi limita la capacità di poter creare delle condizioni per un futuro migliore. Ben altre, Ben altre, quindi, devono essere - a mio modo di vedere - le necessità del Paese e ben altro avrebbe dovuto essere l'utilizzo di questo *extra* gettito.

questa manovra fiscale non va nella direzione necessaria per il nostro Paese in questo particolare momento. Queste che ho testé citato sono le misure proposte dalla Casa delle libertà e, guarda caso, sono proprio le stesse indicazioni che vengono dalla Banca d'Italia, dal Fondo monetario internazionale e dall'Unione Europea. La manovra di questo Governo è negativa per il Paese e deriva

inutilmente le grande energie che il popolo italiano ha messo a disposizione anche attraverso un aggravio della pressione fiscale. Purtroppo, esprimo un parere estremamente negativo su questa manovra e mi auguro che cali il più presto possibile il sipario su questa compagine che non fa bene al Paese. onorevole rappresentante del Governo, colleghi, nelle settimane scorse, abbiamo più volte discusso, in questa stessa Aula, della politica fiscale del Governo, a partire da talune forzature, come il dibattito sul generale Speciale. Insieme ad altri colleghi, anch'io avevo sostenuto allora come la sollecitazione ad affrontare le mozioni presentate al riguardo dai Gruppi di opposizione fosse strumentale ed esse fossero volte più a mettere in discussione una politica che a porre una questione istituzionale. Ho voluto ripartire da lì perché oggi abbiamo un'ulteriore conferma di quella strumentalità e ci è data un'altra occasione per misurare gli effetti tangibili di una redistribuzione delle risorse,

che si aggiungono ai 7,5 miliardi di euro di cui al decreto di agosto, rappresentano il segno di come la lotta all'evasione fiscale sia un aspetto fondamentale della politica del Governo dell'Unione, non solo dal punto di vista della finanza pubblica, diretta alla crescita del Paese e alla giustizia sociale, ma anche dal punto di vista del rafforzamento dell'etica e del senso dello Stato. Questa è la via limpida che abbiamo intrapreso e che rivendichiamo: non più tasse, ma tasse eque, pagate da tutti e rigorosamente utilizzate. In questa politica di redistribuzione abbiamo scelto di dare priorità a interventi di grande valore sociale: nel precedente decreto di agosto abbiamo dato un segno di risarcimento sociale a quei milioni di pensionati che, dopo una vita di lavoro, ricevono poche centinaia di euro al mese. Con questo nuovo intervento, affrontiamo la condizione degli incapienti, di chi ha un reddito talmente basso da non godere di nessun e cominciamo ad aggredire il problema della casa che tanto pesantemente grava, quasi a divorarli, sui redditi di molte famiglie. Accanto all'attenzione per i problemi e le necessità dei più deboli, c'è nel provvedimento una nuova sensibilità verso il tema del sapere e della conoscenza che voglio sottolineare con particolare soddisfazione. Si pensi, ad esempio, alla scelta di aumentare di 150 milioni di euro i fondi disponibili per l'innalzamento dell'obbligo d'istruzione disposto dalla legge finanziaria per il 2007, bloccando peraltro l'operatività della clausola di salvaguardia prevista in quella sede, con l'effetto di rallentare il processo di riduzione del personale scolastico. Congelare la clausola di salvaguardia è una scelta chiara che dà un segno utile a quel mondo della scuola, rispetto al quale crescono, da parte delle società, le aspettative e le domande. Rafforzare la disponibilità economica per l'obbligo scolastico può essere la strada per costruire la scuola di tutte e di tutti che, con l'innalzamento dell'obbligo, vogliamo realizzare. Sarà così se la maggior parte delle risorse andranno ad eliminare quella che è una vera e propria tassa occulta: i libri di testo. È di queste settimane la notizia che anche l'Autorità per la concorrenza ha avviato un'indagine in materia e noi possiamo fare la nostra parte. La gratuità dei libri sarebbe il primo intervento per il diritto allo studio a doversi accompagnare all'innalzamento dell'obbligo scolastico. Altro impegno positivo è quello che consente di sbloccare i fondi per la ricerca scientifica, affidando al Ministero dell'università la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica Eravamo ormai di fronte ad una sofferenza del sistema universitario e degli enti di ricerca che ora potrà essere superato. Siamo allora di fronte ad un intervento utile dal punto di vista sociale, ma anche significativo in termini di sviluppo e crescita del Paese. È nostra convinzione che una società più forte dal punto di vista della cultura e della conoscenza non solo contribuisce alla costruzione di una comunità più equa e coesa, ma anche ad affermare nuove opportunità di sviluppo e di crescita. Cultura e conoscenza significa anche consapevolezza della propria storia. Sull'investimento per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia abbiamo sentito in questi giorni qualche perplessità: sarà compito del Governo fugare tali riserve informando il Parlamento delle iniziative programmate per tali celebrazioni. Nel complesso mi pare un'idea molto valida, perché costruire una forte comunità nazionale, consapevole della propria storia, è un passaggio indifferibile per costruire futuro e speranza. Nella spedizione dei Mille prima e nell'unificazione nazionale poi, noi troviamo il seme che farà poi germogliare la Repubblica dopo la triste parentesi del fascismo. È solo in quel cammino storico che possiamo trovare un futuro, tanto più in una fase convulsa come quella presente. Non si tratta di fare della vuota retorica, ma di ancorarsi a forti e condivisi momenti che hanno sedimentato quello che poi è diventato il nostro Paese. Per questo, sommessamente, abbiamo sollevato la necessità che nella celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che si prepara oggi, la scuola abbia un ruolo importante e primario. Solo la scuola è il luogo della trasmissione del passato alle future generazioni, e da lì dobbiamo ripartire. Nelle fredde cifre dello stanziamento, noi vogliamo leggere un messaggio. La responsabilità di ciascuno, nella propria funzione chiamato, fosse anche nel pagare le tasse, è ciò che consente di riaffermare la nostra comune storia, di progettare un cammino condiviso, di stare vicino a chi è più debole.

Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il nome di Alexander Jonas non dirà nulla alla maggior parte dei colleghi e a tanti nostri concittadini. Così come pochi hanno soffermato la propria attenzione sul piccolo Francesco: si tratta di due morti, uno a soli 2 mesi, a Roma, l'altro a 61 anni, a Trieste, per il primo freddo di questi giorni. Così come a molti i nomi di Giuliano Nascimbeni, di 47 anni, morto nella falegnameria in cui lavorava in Provincia di Padova, e quello di Michele Cozzolino, di 31 anni, colpito da un tubo in una centrale ENEL, non dicono nulla: non sono che gli ultimi nomi della strage che ogni giorno si compie nei cantieri e nei posti di lavoro. Non si può nel 2007 morire per lavorare; non si può morire perché si è cittadini slovacchi e si dorme all'addiaccio; soprattutto, non si può morire a 2 mesi - ripeto, a 2 mesi - perché si e si è costretti a vivere accampati lungo il Tevere, con due genitori poco più che bambini. Inizio da qui il mio intervento sul decreto-legge oggi in discussione e sulla manovra di bilancio, perché è anche per queste persone, per evitare questi gravissimi e altri problemi forse meno gravi, ma più ampi, che colpiscono tante persone e tante famiglie che siamo stati chiamati a governare. È anche per loro e per prevenire i drammi della solitudine, della povertà, dell'iniquità della distribuzione delle risorse, per aiutare il nostro Paese a imboccare una strada di sviluppo che sia anche di uguaglianza, che oggi ci accingiamo a lavorare alla manovra finanziaria. È perché nessuno più debba morire in fabbrica, nessuno più debba non avere una casa, non avere diritto all'infanzia e ad essere considerato un cittadino in sé, anche a soli 2 mesi (e godere, quindi, di uguali diritti di tutti gli altri coetanei, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla condizione sociale dei genitori); è perché, in un Paese sviluppato e ricco come il nostro, dobbiamo avere tra i primi impegni quello di sconfiggere la povertà; è perché il diritto alla salute sia garantito a tutti attraverso un sistema pubblico, universalistico e solidale che consideriamo una priorità la lotta all'evasione fiscale e l'utilizzo equo delle risorse. Così Rifondazione Comunista e la sinistra di Governo salutano con interesse e partecipazione la novità di questa manovra 2008-2010, che è l'avviamento della strategia di redistribuzione sociale. Finalmente, in questo decreto collegato alla finanziaria è prevista la destinazione di 5,9 miliardi provenienti dalla lotta all'evasione fiscale, di cui circa 4 miliardi sono impegnati per iniziative sociali a vantaggio dei ceti più deboli. Questa finanziaria, infatti, non è semplicemente lo strumento per risistemare i conti, ma un'occasione per dare all'Italia una nuova direzione nella politica economica e nell'uso della spesa pubblica. Insomma, oserei dire che in questa finanziaria, che purtroppo continua ad essere uno strumento un po' farraginoso e oscuro anche per chi, come me, è ormai alla sua ennesima finanziaria (figuriamoci per il cittadino elettore), sta pian piano emergendo un'anima. Davvero - lo consiglio caldamente al Governo, e mi sembra che abbiamo timidamente iniziato a percorrere questa strada - la prima cosa da fare sarebbe quella di rendere più semplice il processo di costruzione e di lettura dei provvedimenti in finanziaria, evitando che diventi un *puzzle* in cui alla fine nessuno è più in grado di raccapezzarsi; probabilmente molti colleghi lo sanno fare meglio di me, ma spesso non si raccapezzano più nemmeno i parlamentari e gli esperti di finanza pubblica. Dico questo senza voler arrivare a citare la famosa cuoca di Lenin, per carità, ma ricordando a tutti noi che una norma finanziaria di più facile lettura, anche per il cittadino e la cittadina qualsiasi, sarebbe un gran bel biglietto da visita di un Governo che intende essere popolare. Signor Presidente, non riuscirò ad

che si inseriscono perfettamente nel solco del programma con il quale il Governo Prodi si è presentato agli elettori e che toccano elementi qualificanti su cui verificare la tenuta della maggioranza. Dopo il corteo di sabato, con il quale tanti cittadini hanno chiesto al Governo che sostengono l'attuazione del programma, siamo determinati più che mai ad andare avanti con il nostro impegno e proponiamo un confronto nel merito su materie che toccano così da vicino la vita delle persone,

Signor Presidente, anche se è pura utopia, avrei gradito che fossero presenti oggi in quest'Aula anche il presidente Prodi, il vice presidente D'Alema e il ministro Amato. Avrei voluto chiedere loro - che rispettivamente solo dieci, nove e otto anni fa sono stati Presidenti del Consiglio di questa Repubblica - come possono rimanere impassibili di fronte ad una decisione che ha azzerato, senza alcuna logica motivazione, la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina; come possono aver preso parte all'annullamento di una loro decisione, assunta collegialmente in tre passati Governi da loro stessi presieduti. Tutto per sottostare al ricatto di una microaggregazione politica, quella rappresentata dai ministri Bianchi e Pecoraro Scanio; una minoranza partitica che, solo per motivare la propria esistenza e per produrre un vero condizionamento politico, ha usato il veto, non su un'opera, ma su un processo di sviluppo del Mezzogiorno. Il ministro Di Pietro, intervenendo il 18 ottobre a Napoli alla conferenza sulle opere pubbliche, ha ribadito: "Il furore ideologico ed antagonista di Verdi e di sinistra, un furore simile ai talebani che distruggono i Buddha, costerà allo Stato 500 milioni di euro". Ma al ministro Di Pietro chiedo: come fa a rimanere ancora seduto negli scranni del Governo e come riesce a convivere con coloro che lui stesso ha definito, giustamente, talebani? Ora, però, con questo decreto-legge collegato alla finanziaria siamo arrivati al momento terminale, al momento delle responsabilità, al momento in cui qualcuno, signor Presidente, dovrà rispondere di danno all'erario. Questo mio intervento sarà sicuramente letto dal presidente della Corte dei conti, quindi, siccome sono convinto che in un organismo istituzionale come la Corte dei conti non alberga nessuna logica di schieramento, questa mia denuncia troverà, ne sono certo, un immediato riscontro. La decisone assunta dal Governo, su proposta del ministro dei trasporti Bianchi, causerà un danno al Paese di oltre 1.460 milioni di euro, non di solo 500 milioni di euro, come ha ricordato il ministro Di Pietro, sono relativi solo alle spese di progettazione ed alle penali da pagare alle imprese. L'importo di 1.460 milioni di euro tiene anche conto del mancato avvio dei lavori diciotto mesi fa e quindi del contestuale aumento di circa il 6 per cento del valore globale iniziale dell'opera e cioè di oltre 360 milioni di euro, sia del mancato utilizzo delle risorse dell'Unione Europea, pari ad almeno 600 milioni di euro 10 per cento del valore dell'opera). Il Governo dimentica, infatti, che l'opera, non solo fa parte del Corridoio 1 (Berlino-Palermo), ma è stata scelta dall'Unione Europea e dal Parlamento europeo come una delle 17 opere essenziali delle reti TEN. Nella scelta di questo Governo di non realizzare il ponte, non si è mai, dico mai, affrontato il tema di questo grave danno, non si è mai giustificata una simile scelta antitetica ad ogni logica di corretta gestione della cosa pubblica. Credevo che, in un consesso istituzionale così elevato come il Parlamento, la forza della ragione vincesse sulla forza dell'ignoranza e dell'arroganza. Ritenevo, signor Presidente, che, prima di cadere nella trappola del più bieco integralismo, il Parlamento potesse far capire al Governo, o almeno ad alcuni suoi membri, quale danno, non quello del breve, ma quello del medio e lungo periodo, si stava arrecando al Paese. Infatti, si è caduti nel più assurdo soggettivismo: quello di ritenere la scelta di realizzare il ponte (una scelta confermata dal consenso di dodici legislature, una scelta condivisa e confermata dal Parlamento europeo) e confermata dal Parlamento europeo) un banale capriccio, una banale rincorsa per lasciare un segno sul territorio e non un'esigenza, quella di dare ai cittadini di un'isola un grado di libertà in più per renderli uguali agli altri cittadini del Paese e dell'Unione Europea. Sì, un folle e maniacale capriccio di chi governava in quel momento il Paese, dimenticando che nell'intera storia della nostra Repubblica la realizzazione del ponte sullo Stretto non ha mai avuto schieramenti democratici ad essa antitetici o contrari. Purtroppo, signor Purtroppo, signor Presidente, sta vincendo la forza dell'ignoranza, una forza governata da due ministri, Bianchi e Pecoraro Scanio; due Ministri che abbiamo sempre trovato tra i sostenitori dei "no TAV", dei "no ponte", dei "no MOSE", dei no a tutto ciò che significa crescita e sviluppo. al ministro Pecoraro Scanio fa comodo un Paese non infrastrutturato, un Paese terzomondista, perché solo in tal modo, attraverso il loro integralismo di sinistra, possono gestire il sottosviluppo. Questa grave ignoranza contiene però, come ho detto prima, una chiara responsabilità oggettiva, che non si limita solo ai due Ministri, ma coinvolge direttamente tutto il Governo e tutte le forze della maggioranza; quelle forze, che non hanno nulla a che fare con un folle integralismo di sinistra, ma che hanno vissuto questa grave decisione, succubi solo di una smodata mania di potere. Dimenticando che quando le minoranze, all'interno di una coalizione di Governo, impongono le proprie decisioni, allora di democratico non rimane nulla. Accanto a questa responsabilità oggettiva, a questa irresponsabile incapacità di misurare i vantaggi e gli svantaggi di una scelta, da addebitare a membri dell'attuale Governo ed in particolare ai ministri Bianchi e Pecoraro Scanio, quali portatori solo di un vergognoso ricatto politico, ritengo debba aggiungersi un'altra responsabilità: quella politica. Una responsabilità, quest'ultima, di chi non è all'interno del Governo o del Parlamento, ma che riveste ruoli altrettanto fondamentali. Mi riferisco, in particolare, ai Presidenti delle Regioni del Mezzogiorno e al sindacato. Mi riferisco a tutti i Presidenti delle Regioni del Mezzogiorno, in quanto nessuno di loro ha preferito, per un attimo, spogliarsi della veste partitica, privarsi della banale logica di schieramento, per rivendicare un interesse condiviso, non solo dal Paese, ma dall'intera Unione Europea. Qualcuno potrebbe dire che, in questo elenco di Presidenti del Mezzogiorno, non può essere annoverato il presidente Cuffaro; senza dubbio, il presidente Cuffaro è stato l'unico che ha condiviso e difeso sempre la realizzazione del ponte, ma mi spiace che abbia accettato la quota delle risorse della società Fintecna destinate alla realizzazione del ponte. Quelle risorse potevano essere utilizzate solo «per investimenti che garantivano un ritorno economico certo». Accettando tali fondi, i due Presidenti delle Regioni Sicilia e Calabria si sono assunti, insieme al Governo, una grave responsabilità: hanno in realtà condiviso una vera «distrazione di fondi». Il presidente Cuffaro non doveva farsi attrarre da questo ridicolo specchietto per le allodole con cui il presidente Prodi ha giocato questa miserevole partita. Accanto ai Presidenti del Mezzogiorno non posso non inserire il sindacato. Va dato atto: il sindacato, da sempre, ha difeso gli interessi del Mezzogiorno, e quindi si rimane sconcertati che, dopo diciotto mesi di Governo, nessuno dei rappresentanti

nell'attuale DPEF, con l'azzeramento del ponte sullo Stretto e degli schemi idrici, si ottiene una percentuale per il Mezzogiorno non superiore al 25 per cento delle risorse della legge obiettivo. In tal modo, il sindacato perderà, nel breve periodo, la propria base, in quanto è venuto meno proprio alla sua primaria missione: quella di garantire davvero lo sviluppo del Mezzogiorno. La sostenibilità istituzionale, signor Presidente, come tutti sappiamo, è la capacità di una legislatura di dare continuità alle scelte assunte nelle passate legislature e, nel caso del ponte, ben sette legislature avevano condiviso formalmente la realizzazione dell'opera; mi spiace doverlo constatare ma, quando ciò non avviene, vuol dire che ci si avvia verso forme irreversibili di crisi della democrazia parlamentare. È una responsabilità che questo Governo e, purtroppo, questa legislatura si assumono, nei confronti non solo delle future generazioni di questo Paese, ma di quelle dell'intera Comunità europea. Nessuno in futuro capirà i motivi, le logiche, gli schieramenti ideologici che hanno portato solo ad un risultato: il fallimento concettuale di una vera rivoluzione socio-economica del nostro Mezzogiorno. Un fallimento prodotto da forze ideologiche assimilabili, come dichiara un Ministro dell'attuale Governo, a quelle dei talebani. Ci rivolgiamo quindi, signor Presidente, ai moderati della maggioranza per ricordare loro che oggi si sta decidendo di togliere a sei milioni di italiani, non un semplice tratto di strada o di ferrovia,

Ci rivolgiamo, ripeto ancora una volta, ai moderati della maggioranza, affinché non si mettano, una volta tanto, allo stesso livello di quella minoranza fanatica, eversiva e devastante per lo sviluppo del Mezzogiorno e per il futuro della gente del Sud. *(Applausi

Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, signori del Governo, penso che una manovra economica di qualsivoglia Governo dovrebbe essere misurata e giudicata sulla base della rispondenza ai bisogni dei cittadini,

di rispondere a taluni dei problemi principali del nostro Paese; certamente non li risolve tutti, ma sicuramente ne affronta alcuni in senso pieno e compiuto.

è stato discusso in quest'Aula più volte e che interessa migliaia di famiglie. È un problema talmente all'ordine del giorno che il Governo, poco tempo fa, è stato costretto a reiterare un provvedimento contro gli sfratti,

la gente non paga l'affitto non perché è particolarmente furba ma perché migliaia di famiglie non sono nella condizione di poterlo pagare. Questo è un dramma sociale che dovrebbe interessare tutti.

rilevano che una parte consistente delle famiglie che pagano l'affitto impegna per esso dal 20 al 50 per cento del proprio reddito. Questa è una situazione assolutamente seria, particolarmente pesante che un Governo non può non prendere in considerazione.

da anni, sul quale da anni si disserta ma su cui poco si è fatto. La domanda è: questo decreto affronta o no questo problema? La risposta è affermativa, e lo dico senza alcuna concessione al fatto che faccio parte, con il mio Gruppo, della maggioranza. Lo affronta, e lo fa in maniera compiuta. 750 milioni di euro sono una cifra molto consistente. È una cifra che da anni non veniva messa in campo per le politiche abitative. Lo affronta, quindi, con un congruo e sostanzioso investimento; lo affronta con un investimento che non è *una tantum*, un investimento che oggi c'è e l'anno prossimo non ci sarà

È del tutto evidente che per quanto ci riguarda noi abbiamo investito molto, ci siamo prodigati e abbiamo operato in questa direzione. È un problema quello della casa che sentiamo particolarmente e, quindi, particolarmente siamo contenti che questa manovra economica

uno dei principali problemi che questo Paese ha avuto e spero non avrà più nel futuro.

Il decreto-legge n. 159, che è parte integrante del disegno di legge finanziaria, contraddice sia nella esposizione sia nei fatti la sua descrizione. Questo provvedimento viene descritto come contenente interventi urgenti in materia economico‑finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale; nei fatti, rappresenta non uno, ma molti passi indietro sulla via dello sviluppo, della ripresa economica, delle prospettive del Paese. Lo contraddice - e si contraddice - in quanto gli interventi previsti non si caratterizzano per la loro incisività, per la loro profondità ed efficacia; al contrario, si caratterizzano per la loro superficialità ed evanescenza. Tutto questo è molto grave, perché, nella particolarissima situazione che vive il nostro Paese, vi sarebbe stato bisogno di tutto, eccetto che di improvvisazione o di interventi a pioggia. Vi sarebbe stato bisogno di una politica ragionata, programmata, proiettata verso il futuro e, se vogliamo, anche comparata con le altre economie internazionali (ad iniziare da quelle europee, rispetto alle quali, giorno dopo giorno,

pertanto di trattare alcuni argomenti e articoli che fanno emergere in maniera lampante le discrasie di questo Esecutivo. Si tratta di discrasie sicuramente di natura politica

si interviene sulle Ferrovie con 235 milioni di euro, quando mi pare di poter affermare (anche alla luce degli ultimi articoli pubblicati su importanti ed autorevolissimi settimanali) che queste non abbiano bisogno di interventi a pioggia, ma innanzi tutto di un esame analitico, preciso e puntuale, delle cause del loro arretramento rispetto ad altre ferrovie europee. Hanno bisogno, quindi, di una programmazione, di una verifica e - se mi si consente di dirlo - anche di una bonifica ambientale nel vero senso della parola. parola. Rispetto alle notizie circolate negli ultimi giorni, infatti, sarebbe forse doveroso e opportuno, da parte del Governo, non rimanere in silenzio, ma cercare di chiarire al Parlamento e alla pubblica opinione la veridicità e la sostenibilità delle gravissime accuse sostanzialmente formulate.

ma con una chicca che sostanzialmente lo contraddistingue, lo caratterizza e lo differenzia rispetto agli altri: la costituzione dell'osservatorio nazionale e di quelli regionali sulle politiche abitative, alla faccia del contenimento dei costi della politica. Invece di pensare, per esempio, alla capacità di incidenza del grosso problema dei mutui *subprime* sull'economia abitativa italiana; invece di verificare che oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, neanche a prezzi stracciati alcune fasce della nostra popolazione sarebbero nelle condizioni di acquistare una casa;

A proposito di contenimento dei cosiddetti costi della politica, si veda l'articolo 36, pomposamente rubricato: "Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità nazionale. 150 milioni di euro a pioggia, quando questa iniziativa si dovrà tenere nel 2011, per cui non costituisce assolutamente materia urgente da inserire all'interno del decreto-legge, anche se capisco - e non è ironia

forse per accontentare qualche forza politica o per tenere buono qualche senatore che potrebbe mettervi nelle condizioni di andar via o - a proposito di edilizia abitativa - di sfrattarvi proprio dall'Aula di Palazzo Madama: questo è l'obiettivo che state cercando di raggiungere? Non credo che sia molto autorevole, prestigioso e credibile passare per il Governo delle mance, perché questo è il Governo delle mance. E una mancia disonorevole a mio avviso costituisce anche quella dei 150 euro dati agli incapienti. Gli incapienti, i poveri non vogliono elemosine, vogliono prospettive di lavoro e di inserimento sociale, vogliono prospettive relative alla possibilità di farsi una famiglia e non delle mance che non servono assolutamente a nulla, anzi suonano a disdoro di chi le riceve, ma soprattutto di chi le dà. In sintesi, quindi, anche questo provvedimento è significativo rispetto all'incapacità di questo Governo di affrontare le più grandi questioni che affliggono il Paese. Pensiamo alle grandi battaglie, come quella del risanamento. Avete dilapidato i vari "tesoretti" senza aver fatto un passo indietro rispetto all'ammontare del debito pubblico. Avete perso la battaglia della crescita. Il nostro Paese è quello che cresce meno in Europa, cresce meno anche rispetto ad alcune economie come quelle dei Paesi dell'Est che nel passato avevamo distanti di molto. Oggi, invece, tutto questo non avviene più. Siete stati sconfitti sul fronte della riduzione della pressione fiscale: ma non è ridicolo dire che siamo al 43 per cento come se fosse una vittoria? E non è ancora più ridicolo (anzi io direi pure patetico) dire che la pressione fiscale diminuirà dello 0,001 entro l'anno prossimo? Avete dilapidato anche il maggiore gettito in termini monetari e finanziari che non è stato il frutto delle vostre battaglie contro l'elusione e l'evasione, ma della virtuosità del precedente Governo. E siete stati sconfitti sul terreno che doveva essere per voi il più privilegiato: l'equità sociale, la difesa e la tutela dei più deboli. Ma soprattutto sarete sconfitti in Parlamento e nel Paese.

signor rappresentante del Governo, alcuni mesi dopo la denuncia dei disastri della finanza pubblica annunciati dalla commissione Faini, incaricata dal ministro Padoa-Schioppa di monitorare i conti pubblici, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, a settembre 2006, annunciava con la relazione previsionale e programmatica che le entrate per il 2007 sarebbero state pari a 434,9 miliardi di euro. Nel settembre 2007, lo stesso documento approvato dal CIPE innalzava le entrate previste a 456,3 miliardi di euro, ossia a una previsione di maggior gettito di 21,4 miliardi di euro. La corsa alle entrate, però, non finiva qui. Con la previsionale approvata il 28 settembre scorso, la notte di approvazione della finanziaria da parte del Governo, il tetto delle entrate si è alzato a 474,5 miliardi di euro. In due anni, tra il 2007 e il 2008, il Governo ha previsto di incassare maggiori tributi per quasi 40 miliardi di euro. A questi valori sono da aggiungere i maggiori contributi sociali per 15,7 miliardi di euro nel 2007, rispetto al 2006, che saliranno però di altri 10 miliardi nel 2008. Questa posta di entrata Berlusconi se la sarebbe potuta sognare. Fortuna che c'è un Governo vicino agli operai e ai precari! Sommando quanto questo Governo ha sottratto al sistema delle imprese e delle famiglie negli anni 2006 e 2007 per destinarlo allo Stato, si arriva alla cifra da capogiro di 65 miliardi di euro. Prodi ha sottratto ricchezza agli italiani per sé e i suoi amici di centro-sinistra per il 4,3 per La metà di queste cifra, infatti, servirà a coprire una maggiore spesa pubblica di 30 miliardi di euro: tanto è cresciuta tra il 2006 e il 2008, che ci accingiamo a prevedere con la finanziaria in esame. Solo una parte di questa entrata stratosferica servirà al risanamento dei conti pubblici. Il comma 4 dell'articolo 1 della finanziaria 2007 stabiliva che, se si fosse registrato un maggior gettito derivante da tributi rispetto alle previsioni, lo si sarebbe dovuto destinare alla riduzione del disavanzo e quindi del debito pubblico. Il successivo comma 5 disponeva che entro il 30 settembre il Governo era tenuto a presentare una relazione dove avrebbe evidenziato quanta parte del maggior gettito tributario era di natura permanente e quanto dovuto all'andamento ciclico dell'economia, quindi a carattere temporaneo: dei due commi, il primo non è stato adempiuto e per il secondo - ci giunge notizia - è stata consegnata la relazione solo qualche ora fa. fa. Il maggior gettito di 18 miliardi di euro è stato in parte destinato al decreto-legge n. 81 dello scorso luglio per 7.403 milioni di euro, in parte al al decreto-legge n. 159 per circa 6 miliardi di euro e per la parte restante destinato alla finanziaria 2008, a causa di questa dissipazione di tesoretti, il disavanzo è cresciuto al 2,5 per cento del PIL nel 2007 e il debito pubblico,

Invece di alleggerire il carico di debiti alle future generazioni lo avete appesantito. È una politica finanziaria da irresponsabili per due motivi: il primo, perché queste risorse tributarie - come vedremo - non sono destinate allo sviluppo, quindi con ricadute positive verso le future generazioni, ma a sostenere richieste volatili a carattere elettoralistico; secondo, perché in uno momento di crescita economica avremmo dovuto utilizzare le maggiori entrate che si determinano e si determineranno per il risanamento, ovvero per gli investimenti, soprattutto se permanenti. contrario le maggiori entrate tributarie derivanti dell'aumento della pressione fiscale - che ha raggiunto la cifra *record* del 43 per cento, pari a quella che si registrò nel 1997, quando l'Italia scelse l'euro,

43,2 per cento - dovevano essere restituite agli italiani, migliorando la quota di reddito destinata al risparmio e ai consumi, per il rilancio dell'economia e della domanda interna in particolare. Ne avrebbero beneficiato famiglie ed imprese, soprattutto i giovani e l'occupazione, combattendo il precariato con politiche reali e non con le mance di Stato a favore di chi versa in stato di bisogno. C'è un proverbio cinese che recita: «Se uno ha fame, non dargli il pesce ma insegnagli a pescare»; voi invece state distribuendo pani e pesci, invece di proporre una decisa politica di riforme, che dia efficienza economica, liberando i mercati da vincoli e da protezioni, che elimini la spesa inutile ed improduttiva, che alleggerisca il costo diretto della burocrazia e quello indiretto degli adempimenti con un forte processo di semplificazione, continuando quell'opera meritoria che anche lei, presidente Baccini, da ministro della funzione pubblica, aveva con successo iniziato. Niente di tutto questo. La riforma dei servizi pubblici locali è al palo, anzi è tornata indietro rispetto alle aperture proposte che anche l'UDC aveva considerato da valutare positivamente. Il federalismo fiscale è al palo anch'esso, con una riduzione degli spazi di responsabilità delle autonomie locali, che oggi lo contestano,

fortemente ipotecata da un rinnovo del contratto 2006/2007 che prevede uno scivolamento verso l'alto delle qualifiche senza merito e senza risultati di produttività. La riforma del *welfare* si è limitata a peggiorare i conti pubblici della previdenza senza preoccuparsi dei disoccupati e della famiglia, che registrano il peggior tasso di incentivi pubblici dell'Unione Europea. Queste misure hanno avuto effetti depressivi sulla nostra economia, soprattutto hanno ridotto la domanda interna, tanto da rivedere al ribasso per il 2007 e il 2008 le stime di crescita previste nella Nota di aggiornamento al Documento di Noi dell'UDC, attraverso il sottoscritto, allora lo denunciammo con decisione. Fummo inascoltati, ma i fatti ora ci danno ragione. Con questo decreto ci si aspettavano, quindi, misure per lo sviluppo. Ce ne sono alcune che vengono spacciate per tali, ma che tali non sono. Il resto è una legge mancia. Che di mancia si tratti lo si deduce dall'elenco delle misure previste: contributi alla rete ferroviaria italiana e all'ANAS; contribuiti a Roma, Milano e Napoli per la metropolitana; contributi per affrontare l'emergenza trasporti sullo stretto di Messina dopo la cancellazione del ponte; contributi a Trenitalia Spa; contributi al Ministero dell'istruzione; contributi in materia di pubblico impiego; contributi all'ONU, per la pace e lo sviluppo, per la Corte internazionale, per le organizzazioni umanitarie, per la distruzione delle armi chimiche in Russia e quant'altro è previsto nella cooperazione internazionale; contributi aggiuntivi al 5 per mille; contributi per l'edilizia residenziale pubblica; contributi per Venezia, per il polo di ricerca Erzelli in Liguria, per i Comuni in dissesto finanziario, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, per i lavoratori socialmente utili della Calabria, per l'ONAOSI, per i ciechi e i sordomuti, per l'ENEA e la Finmeccanica, per i talassemici, per le zone di confine, per il 150° anniversario dell'Unità nazionale e via di discorrendo. Siete stati timidi e con le braccia corte sugli incapienti. Avete destinato loro appena 150 euro l'anno e per il solo 2007, come se per il 2008 diventassero ricchi. Gli incapienti sono coloro che non percepiscono i vantaggi delle deduzioni e delle detrazioni fiscali perché non hanno reddito, ovvero il reddito è così basso che non sono tassabili e quindi non hanno sgravi fiscali. Sono 12 milioni e mezzo di persone. Ebbene, per costoro solo 12 euro al mese, collega Bonadonna, mezzo chilo di pane ogni due giorni, e solo per il 2007. Niente per il 2008. Forse avete reintrodotto la tessera. Eppure è uno dei pezzi forti del vostro programma, insieme a quello dei non autosufficienti di cui vi siete dimenticati anche in finanziaria. Anche a questi compagni comunisti avete girato le spalle per qualche Ministero e Sottosegretario in più? Vi siete convertiti alla grande editoria, finanziando senza pudore i grandi gruppi editoriali della FIAT, della Confindustria, dei palazzinari, persino di Berlusconi, senza battere ciglio. Avete votato all'unanimità, insieme ad altri alleati del centro-destra, contro il mio emendamento di riduzione del 50 per cento dei contributi all'editoria e soprattutto alla grande editoria. È questo il prezzo del potere? Che questo prezzo sia il prezzo, lo avete dimostrato votando contro l'emendamento del collega Calderoli alla Nota di aggiornamento al DPEF 2007 sulla riduzione dei Ministri e dei Sottosegretari. Spero che i senatori Bordon e Manzione ci riprovino tra qualche giorno, così vedrò come si muove il pensiero e la mano del senatore Salvi, di Rifondazione Comunista e dei dipietristi. A parte altre considerazioni politiche, né sul disegno di legge finanziaria per il 2008 ci sono sgravi fiscali sul lavoro, soprattutto sui redditi più bassi; non ci sono misure per la conciliazione tra lavoro e impegni familiari, come il famoso annunciato piano piano per gli asili nido e gli incentivi alle madri lavoratrici facevano prevedere, per alzare il tasso di occupazione delle donne secondo le indicazioni dell'Agenda di Lisbona. Queste misure, che sono misure per lo sviluppo, sono state sacrificate per gli sgravi ICI che hanno un effetto limitato sulla domanda interna. È mancato il coraggio di essere riformisti o riformatori; è mancata la capacità di essere governanti e uomini di Stato. Per queste ragioni

la cartina di tornasole della miseria politica, morale e programmatica del Governo, del Presidente del Consiglio e di un Ministro presunto economista ma in realtà banchiere.

Per l'equità sociale in tutto sono 750 milioni di euro; ricordo che il Governo Berlusconi, con due interventi in materia fiscale, prese provvedimenti per 14 miliardi di euro. Quindi questo Governo di sinistra, sostenuto da Rifondazione Comunista e anche dai movimenti, si va manifestando ogni giorno come il Governo della speculazione, dei banchieri e delle oligarchie.

sono state per 16,8 miliardi di euro; con il Governo Berlusconi e con il ministro Tremonti le risorse evase accertate ammontavano a 19,4 miliardi di euro. euro. Spendete i soldi ma non siete in grado di scovare gli evasori. Non siete in grado neanche di scovare gli evasori totali, perché siete stati capaci nel 2006 di scovarne meno di quanti furono nel 2005. Siete degli imbroglioni:

Avete letteralmente rubato 4 miliardi di euro ai Co.Co.Co., ai collaboratori coordinati e continuativi, per coprire parte della spesa di 10 miliardi necessaria per mantenere

l'età pensionabile. Spenderete 10 miliardi di euro per la scalinata di Prodi. Quei 10 miliardi di euro potevano essere utilizzati per assicurare una rete di protezione sociale per i precari, per quegli italiani che guadagnano 1.000-1.200 euro al mese. Gli italiani che guadagnano 1.000-1.200 euro al mese e che tirano a campare voi li provocate li provocate con un provvedimento per l'equità sociale, annunciato spagnolescamente da questo disegno di legge, prevedendo 13 euro al mese per ogni nucleo familiare, uno sconto dell'ICI di 10-16 euro al mese, un *bonus* per gli incapienti di 12 euro al mese, mese, un incentivo di 3 euro e mezzo al mese per i bambini che vanno in palestra o vanno a nuotare in piscina. Non vi vergognate? Questo è un Governo inutile e dannoso. È un Governo commissariato dalla grande finanza. È un Governo che non batte ciglio di fronte a un ragazzotto di 40 anni - tale banchiere Arpe che viene liquidato da Geronzi, nei cui confronti si è comportato da vero e proprio estorsore in doppiopetto. Questo Arpe, inoltre, era un allievo del professor Prodi, il quale, come tutti sanno, è uno che vive modestamente, pur avendo guadagnato nei cinque anni di presenza a Bruxelles quanto guadagnano in una vita i 2.000-2.500 metalmeccanici di Torino.

banche. Portate avanti una finanza allegra che incrementa la spesa pubblica primaria. Con il decreto di luglio e con questo in

che questo Paese ha avuto negli ultimi 35 anni. La spesa pubblica ormai è un cancro per questo Paese, ma perché essa cresce con voi? Cresce Cresce per un motivo semplicissimo: questo è un Governo che opera la politica del voto di scambio di massa.

affatto pesanti, anche se possono infastidire il Governo. In quest'Aula, nella precedente legislatura, non solo venivano usati termini estremamente pesanti, ma si minacciava addirittura di aggredire il presidente del Senato, il senatore Pera.

da incapaci. Ha tentato di difendere gli interessi dei grandi sistemi bancari, ha venduto l'anima e il Paese alla grande speculazione, ai grandi gruppi parassitari a quelle che un tempo venivano definite, nel gergo di Giolitti, le mafie meridionali, quelle che meritavano l'interdizione di un uomo come Salvemini. Non a caso, quando